Grazie,

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, noi sosteniamo l'emendamento 3.12 che propone una buonuscita compensatoria per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non si vedono rinnovato il contratto a tempo indeterminato.

Poiché avete reintrodotto le causali, ad esempio un lavoratore o una lavoratrice impiegata in un'azienda dolciaria per produrre panettoni a Natale

Il mio collega, senatore Paragone può fare tutta la propaganda che vuole in quest'Aula, ma succederà questo, perché questa è la verità dei fatti. Quando ieri dicevo che queste norme ledono il principio di realtà intendevo esattamente questo. tentiamo ancora in quest'Aula, ministro Di Maio, di pensare che voi possiate ravvedervi, ma lo diranno i fatti, lo diranno i cittadini e le cittadine, i lavoratori e le lavoratrici che si troveranno da oggi

Grazie,

Se fosse vero - e non lo è - leggendo il provvedimento che stiamo esaminando verrebbe da dire che siamo stati proprio bravi, perché in questo decreto - qui sì - dei lavoratori e dei loro problemi non c'è neanche l'ombra. È invisibile il tema della qualità del lavoro e di come si incentiva il lavoro stabile. È invisibile il tema delle competenze e della formazione. È invisibile il tema salariale, dei bassi salari e dell'equità nei trattamenti retributivi. Sono invisibili quei milioni di lavoratori a basso reddito, che aspettano una paga onesta per un lavoro onesto e non un reddito per non lavorare. Questo decreto-legge è una *fake news*. Si dice di fare come in Europa, portando il tempo determinato a ventiquattro mesi, ma si viola una direttiva comunitaria sulla somministrazione, come ha spiegato la senatrice Parente. Si dice di avere a cuore il lavoro, ma poi si fa una norma transitoria pasticciata, che sta creando il caos tra imprese e lavoratori, con il risultato di distruggere posti di lavoro. Si dice di introdurre nuovi incentivi per l'assunzione dei giovani e per la trasformazione del tempo determinato a indeterminato, senza dire che quegli incentivi esistono già, perché li hanno messi i Governi a guida del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E in questo decreto-legge ci si limita a estenderli marginalmente, senza peraltro mai citarli nel testo normativo. Attenzione, lo dico tra parentesi, ma questa fissazione di segnare l'anno zero con la propria presa del potere, cancellando tutto quello che viene prima non ha mai portato bene nella storia. A furia di voler cancellare tutto, si può finire per cancellare anche decenni di progresso scientifico, come avvenuto in quest'Aula sui vaccini. Si dice, ancora, di licenziare il *jobs act*, ma non si toccano neanche i cardini di quella riforma. Restano gli ammortizzatori sociali, restano le nuove linee tracciate tra lavoro subordinato e autonomo, resta l'impianto di politiche attive e resta il contratto a tutele crescenti, che non viene abolito da questo intervento, tanto che la maggioranza ha votato contro un emendamento volto a reintrodurre l'articolo 18; emendamento - questo sì - visibile. Chi se l'è perso pur votandolo può ricercarlo nei verbali. Smettete di dire che siete contro il *jobs act*, perché l'avete appena votato. le *fake news* ci sono sempre state: si chiamavano propaganda politica. I grandi partiti di massa hanno sempre combattuto per l'egemonia culturale, propagandando la loro visione della realtà e della storia, ma sapevano distinguere tra il momento in cui si devono vendere le proprie scelte, anche con la propaganda, e il momento in cui si devono prendere quelle scelte, impedendo che la propria propaganda offuschi il momento decisionale, producendo effetti collaterali perversi sulla vita delle persone. Questo senso di responsabilità istituzionale e questa capacità di distinguere tra propaganda e momento della scelta in questo decreto è del tutto assente. Per questo è una *fake news* e purtroppo la realtà Grazie, Grazie, della maggioranza, che non ha voluto migliorare una virgola o entrare nel merito delle nostre proposte. Abbiamo fatto proposte sul lavoro stabile, su come ridurre il cuneo contributivo sul tempo indeterminato (il Ministro ieri, in replica, ha detto che il Governo intende farlo e vedremo nella legge di bilancio se ci saranno i soldi) ed è per questo che mettono una norma transitoria al 31 ottobre. Vorrei allora dirle, signor Ministro, che quella norma transitoria è un refuso: avreste dovuto metterla al 31 dicembre. E avremmo potuto migliorare quel refuso e i tanti pasticci presenti in questo decreto-legge se qualcuno non avesse avuto l'ansia di sbandierare risultati che non ci sono e avesse lasciato a questo Parlamento e a questo Senato il tempo di lavorare. Le altre proposte che abbiamo illustrato erano quelle di una buonuscita compensatoria, di un salario minimo, di estendere la disciplina del lavoro subordinato ai finti lavoratori autonomi organizzati mediante piattaforme e stringere le false cooperative, perché per noi il vero precariato si annida in queste fragilità del mercato del lavoro, non negli interventi manifesto di questo decreto-legge. Non c'è stato permesso di parlare di queste cose. Continueremo Continueremo a portarle avanti nel Paese e per il Paese.

sia per i lavoratori in somministrazione che per i lavoratori a tempo determinato e noi, di fatto, in questo decreto-legge rispettiamo tale direttiva. Riguardo agli incentivi, all'interno del decreto-legge curiamo in modo particolare il disagio e la disoccupazione che hanno colpito le fasce giovanili nel nostro Paese

in caso di conciliazione e abbiamo portato l'offerta di conciliazione, che prima era da 2 a 18 mensilità, a da 3 a 27 Riguardo poi ad altri interventi migliorativi rispetto a precedenti normative, anche nei successivi articoli, ad esempio con riferimento ai centri per l'impiego, iniziamo

anche in Italia i servizi per l'impiego funzionino e queste - consentitemi di dire - sono le fondamenta per una buona riforma del lavoro che, con il decreto dignità, muove i primi passi.

come evidenziano i dati, è aumentato in percentuale importante, troppo importante, in Italia e che forse siamo uno dei Paesi in cui c'è stato e c'è più precariato,

Parto da una riflessione fatta dal professor Massimo D'Antona in un suo saggio, secondo il quale la questione centrale per il futuro del diritto del lavoro è quella di equilibrare le protezioni del lavoro oltre la subordinazione, senza rinunciare alla tutela specifica di quest'ultima. L'urgenza di apprestare un nuovo principio regolatore attiene alla dimensione politica della partita. questo mi sarei aspettato da un Governo del cambiamento e non questa specie di ossessione luddista di distruggere tutto quanto fatto dai Governi Renzi e Gentiloni

e l'obbligazione che lei, ministro Di Maio, ha contratto con il Paese si è trasformata in una prestazione impossibile e, con questo provvedimento, diventa tutto più chiaro, soprattutto per i lavoratori.

questo emendamento, con tutte le proposte inanellate dal collega Nannicini, emerge in modo chiaro, univoco e non equivoco la proposta politica del Partito Democratico, che è legittima

Sappiamo e siamo consapevoli che ogni Governo che si è insediato, nella storia della Repubblica, ha avuto l'obiettivo

è quale terapia si va a somministrare: il paziente si rivolge a un medico, che gli somministra una terapia; un altro medico gli somministra un altro tipo di terapia; a distanza di tempo si capirà - a volte, non sempre - se c'è una terapia sbagliata. Noi siamo convinti, legittimamente, a differenza vostra, che la terapia contenuta nel decreto dignità sia

Quanto alla forma, che in politica è sostanza, ci sono due forze politiche che hanno fatto - e si sono contraddistinte, per la loro relativa cifra - delle battaglie politiche negli ultimi anni

a leggere anche una sola pagina del contratto gialloverde: sul tema del lavoro, secondo noi, ci sono delle incongruenze o, comunque, niente o poco o solo un alito è stato fatto, che trova scarsa forma e concretezza nel decreto-legge dignità. Anzi, ci sono delle sostanziali contraddizioni. E qual è l'altra contraddizione? Che fate un decreto di urgenza e nel momento in cui un Governo propone un'urgenza su alcuni temi, mi viene spontaneo

non devo farla io la lettura e non dovete farla voi, la devono fare gli italiani. Ministro Di Maio, sa quando si scoprirà chi ha ragione o torto, al di là della danza di natura dialettica all'interno di quest'Aula? Tra sei mesi ci sarà una sentenza inoppugnabile: ci saranno i dati e quei dati sul lavoro e sull'occupazione dovranno essere comparati con i dati dell'occupazione e della qualità dell'occupazione al 4 marzo. In quel momento, con il monitoraggio, gli italiani vedranno chi ha ragione e chi ha torto. Oggi, noi siamo all'opposizione e voi avete il potere. Però, sfortunatamente per gli italiani e con preoccupazione per noi, quella sarà la sentenza.

sostengo questo emendamento che è teso a contrastare le false cooperative e ci serve, in fondo, colleghi, per ragionare su quello che stiamo facendo. Lei, Vice Presidente, ha già dichiarato più volte che occorre intervenire contro le false cooperative

avete proceduto peggio che se aveste posto la fiducia, perché nelle Commissioni non avete consentito che ci fosse una discussione reale. Abbiamo fatto una finzione: nelle Commissioni non si è discusso nemmeno dei pareri dell'Ufficio tecnico del bilancio, che ha sollevato questioni cui il Governo non ha risposto: non una risposta. Alla faccia del rispetto del Parlamento!

e, in effetti, avevamo tutti accettato il monitoraggio di questa legge, che evidentemente andava fatto ma, per la verità, il MoVimento 5 Stelle si è opposto perché non c'era nel contratto.

Bisogna combattere questo fenomeno e l'emendamento 3-*bis*.3, in effetti, fa riferimento ad un'organizzazione pensata all'interno dei centri per l'impiego, là dove evidentemente bisogna istituire un programma di prenotazione, assunzione e riassunzione. Questo emendamento - lo dico, sempre per il tramite del Presidente, al Governo e al Ministro - ha riportato il parere favorevole della Commissione. Non mi trattengo quindi su un fenomeno che conosciamo molto bene, non ci sono i tempi: lo faremo in Commissione, quando il Ministro sarà presente a parlare non con i tempi contingentati, che non ci piacciono, ma con la disponibilità che meritano questi argomenti. *(Applausi dal Gruppo

per affrontare la questione del precariato all'interno della scuola. Chiunque abbia messo mano, in tutti questi anni, al sistema di istruzione italiano, in realtà non ha affrontato quella che è diventata una vera e propria piaga del sistema e che, ovviamente, lo indebolisce. Stiamo parlando di vicende che vanno

Grazie,

- leggo dal testo - trasformati «in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019». Quindi è chiaro, certificato e scritto da loro che il decreto-legge licenzia

e le sentenze si rispettano sia quando si è maggioranza che quando si è opposizione. So che voi rimpiangete un sacco quella bella opposizione con *l'hashtag*

applicata anche a questo caso. Così potrete spiegare ai maestri perché non avete avuto voglia di utilizzarlo e dal 30 giugno li lascerete a casa. Vi abbiamo chiesto anche un'altra cosa, perché abbiamo capito che avete inteso finalmente, a distanza di tre anni, l'utilità della legge n. 107 del 2015, tanto che all'interno di una delle vostre relazioni tecniche scrivete

della senatrice Ronzulli).* Infatti, se voi non metterete in maniera chiara una data certa per i concorsi, ricreerete un'altra graduatoria che quel precariato lo aumenterà.

laureati in scienze della formazione primaria possono partecipare solo se hanno ventiquattro mesi di servizio e non vi rendete conto che i laureati in scienze della formazione primaria, con questa norma che voi create, a questo punto non potranno più lavorare. Non solo: non vi rendete neanche conto di come è composta la facoltà di scienze della formazione primaria, che già prevede al suo interno il tirocinio per questi studenti, i quali sono quindi pronti ad entrare in classe. Ce lo dovete spiegare voi. Ci dovete spiegare anche un'altra cosa: perché avete bocciato e espresso il parere contrario a tutti i nostri emendamenti che potenziano i posti al Sud? Ministro, vi abbiamo chiesto 6.000 6.000 posti all'anno. Non vi chiediamo di arrivare ai livelli del Governo Renzi, che in un anno ne ha assunti 140.000. *(Applausi

stregoni sulla pelle degli italiani e dei bambini. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su una realtà molto difficile. Noi abbiamo ereditato una situazione complessa e, come tutte le realtà complesse, non hanno soluzioni semplici. Ciò è noto a tutti ed è chiaro. Non saranno certo, purtroppo, ahimè, degli emendamenti a un decreto-legge a poter risolvere tutte le situazioni della scuola di cui siamo consapevoli, anche perché molti di noi in prima persona hanno vissuto le conseguenze della buona scuola.

#Io sto con le maestre proprio perché, in virtù della necessità di rispettare la sentenza, abbiamo trovato una soluzione che consiste, intanto, nel poter mantenere la continuità scolastica e quindi permettere il prossimo anno a queste maestre di restare al loro posto, con i loro ragazzi. Nel frattempo, si sta pensando a un concorso straordinario, che permetta a queste maestre di rientrare dalla porta principale nella scuola dove hanno diritto di tornare. Il concorso straordinario, ovviamente, tutela ed è necessario per una parte di insegnanti, quelli che, appunto, sono i precari. Per cui, i laureati in scienze della formazione, che, come ben sappiamo, hanno fatto nel loro percorso di studi 500 ore di tirocinio, non sono paragonabili a docenti

Proprio per questo seguiranno dei concorsi ordinari biennali nei quali troveranno posto e collocazione i nostri giovani laureati, che hanno anche loro diritto di entrare nel mondo del lavoro. Pertanto questo è un decreto-legge che non risolverà le situazioni della scuola nel suo complesso. Lo sappiamo. Questo è un decreto-legge con cui abbiamo cercato di dare risposta a un'urgenza che abbiamo ereditato e di cui ci facciamo carico senza problemi.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, a che ordine dei lavori si riferisce? Presidente, so benissimo di essere spesso indisciplinato e lei fa bene a rivolgersi verso di me quando, com'è capitato poco fa, ho urlato nei confronti di una collega. Però, mi aspetto da lei lo stesso identico trattamento quando accade il contrario. Siccome la mia collega Malpezzi è intervenuta con parecchi colleghi che hanno sbraitato contro di lei e urlato di tutto e lei non ha detto una parola, le chiederei di utilizzare lo stesso identico trattamento per tutti i senatori in questa Assemblea. Capita troppo spesso che chi presiede abbia verso i colleghi e componenti del Partito Democratico un atteggiamento più ostile rispetto agli altri. Per cui io la richiamo a un atteggiamento che sia più uniforme per tutti i senatori.

Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire anche per illustrare tutti gli emendamenti presentati da Fratelli l'Italia, ma non mi ha visto. Quindi colgo l'occasione adesso,

Relativamente al problema causato dalla sentenza del Consiglio di Stato, ricordo a tutti noi che essa riguarda circa 50.000 maestre di scuola materna ed elementare, iscritte nelle graduatorie a esaurimento con riserva, e circa 7.000 insegnanti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva, dopo aver superato l'anno di prova. Fratelli d'Italia ritiene necessario che si intervenga con una soluzione definitiva e adeguata, non con una soluzione tampone come quella prevista dal decreto-legge, che purtroppo mette solo una pezza provvisoria, rimandando la soluzione del problema che, secondo noi, deve essere al contempo anche rispettosa degli oltre 100.000 insegnanti laureati in Scienze della formazione primaria. La verità - e qui mi meraviglio dell'atteggiamento dei colleghi senatori del PD - è che tutto questo è stato creato dalla buona scuola. La responsabilità è la vostra. ha creato solo una guerra fra poveri, non risolvendo i veri problemi strutturali e organizzativi del comparto della scuola. È giusto anche assumerci assumerci ognuno le proprie responsabilità. Ma, nel rispetto delle responsabilità, è paradossale che anche voi, signori del Governo, colleghi della maggioranza, non vogliate dare una risposta certa a questo problema e non vogliate riconoscere la professionalità di chi per anni ha insegnato ai nostri figli. Cosa facciamo, allora? Facciamo rifare le elementari a tutti i ragazzi allievi di quelle maestre che oggi non hanno il riconoscimento della loro professionalità? (Questa chiaramente è solo una provocazione.) Anche in questo caso, rispetto all'enfasi con cui il Ministro ha annunciato il provvedimento, con rispetto ovviamente dei docenti che qualche beneficio potranno pure avere, verrebbe da dire che c'è stato molto rumore per quasi nulla, non avendo risolto il problema alla sua radice. Gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia vanno nella direzione di sanare questa situazione. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti con i quali chiediamo di confermare tutti i docenti assunti che hanno già superato l'anno di prova; oppure a quelli con cui chiediamo la proroga di due anni delle GAE e l'inserimento nelle GAE

In questo caso sono precari di Stato, sono precari creati direttamente da noi, dal Governo. In questa direzione dobbiamo rendere la dignità alle maestre e ai precari della scuola. Infine, vorrei ricordare che non possiamo nasconderci - lo dico ai colleghi di maggioranza - dietro alle sentenze, perché la magistratura applica le leggi, ma noi le facciamo. Quindi, se abbiamo la volontà politica, possiamo risolvere il problema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ci tenevo a presenziare le ragioni dell'emendamento 4.38, e a leggervi un messaggio arrivato da una di queste insegnanti «Mentre sgrano il rosario virtuale e rimugino su tutti gli incontri fatti, sui discorsi, le paure e le lacrime e su tutta la vita che mi scorre davanti e sul futuro di cui mi vogliono privare, sento un macigno sul petto. Penso alla famiglia lontana: sacrifici e ancora lacrime. Lo sconforto è misto a quell'esile filo di speranza, che non mi vuole proprio abbandonare. Un filo di speranza testardo, come me. Ripenso alle troppe ingiustizie e sento la vita appesa ad un filo

Signor Presidente, colleghi, parliamo della disciplina del concorso straordinario per la copertura di posti per la scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, che sarà bandito e riservato esclusivamente ai docenti che negli ultimi otto anni scolastici abbiano svolto almeno due anni di servizio nella sola scuola

ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione italiana, della legge n. 62 del 2000 e di svariate risoluzioni europee. Forse a questo Governo sfugge (e peggio sarebbe se lo si fosse fatto scientemente) che i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria esclusi dal dettato della legge hanno gli stessi titoli dei colleghi della scuola statale. Forse a questo Governo sfugge che gli alunni delle scuole dove insegnano questi docenti conseguono un titolo equipollente e sono ammessi al grado successivo senza esame di idoneità. Come si possono contraddire questi aspetti escludendo i docenti della scuola paritaria? Forse a questo Governo sfugge che la formulazione attuale va nella direzione di escludere (e quindi discriminare) una categoria importante, i 200.000 docenti che operano oggi nella scuola pubblica paritaria. Forse a questo Governo sfugge che questo è un limite per la libertà professionale ed è una vera e propria discriminazione professionale. Aggiungo che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una docente per il riconoscimento degli anni di servizio svolti nella scuola paritaria e quindi, ai sensi di questo pronunciamento, è inammissibile un dettato che discrimini i docenti che svolgono servizio presso una delle due gambe del sistema pubblico pubblico italiano. È una esclusione che penalizza una categoria di docenti che certamente avranno titolo di fare una marea di ricorsi, che ignora che il sistema scolastico di un Paese di diritto come l'Italia deve essere pluralista nella gestione di un servizio pubblico, come avviene anche nella sanità,

sa molto bene di cosa parla, perché ha partecipato anche lui al concorso del 2011. La legge n. 107 del 2017 è stata una palese iniquità per tutta la classe docente. Noi campani, con commissioni non solo indagate ma addirittura imputate, con commissioni destituite durante lo svolgimento delle prove orali dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, siamo ancora qui ad aspettare che si faccia giustizia. Oggi, approvando questi emendamenti, possiamo finalmente ripristinare una situazione di equilibrio e di serenità. Ecco perché annuncio il mio voto favorevole e mi auguro che lo facciano anche il Governo e questa Assemblea. Grazie,

e propongo di trasformare l'emendamento 5.0.1 in ordine del giorno.

Presidente, ringrazio anche i rappresentanti del Governo che sono presenti. Sono contento che si sia trattenuto oggi anche il ministro Di Maio per seguire questa parte del lavoro di competenza dell'Assemblea. In quest'Aula è stato seduto un importante senatore abruzzese, Silvio Spaventa; è stato un senatore che ha fondato gran parte del diritto amministrativo e ha spiegato a generazioni di studiosi del diritto e anche a generazioni di politici e decisori pubblici che la delibera di un Parlamento non è sicuro che diventi, con immediatezza, con facilità, norma nell'ordinamento. Nel senso che la delibera dell'Assemblea legislativa può anche essere guidata da buone intenzioni, ma poi può avere difficoltà a diventare realtà effettiva, ad avere capacità di miglioramento della realtà effettiva. Penso che la norma del decreto-legge riguardante la dignità delle imprese per quanto concerne il rispetto nei confronti del lavoratore, del territorio, dell'ordinamento nazionale, cioè quella norma che stabilisce delle sanzioni,

una norma funzionante del gennaio del 2014, che stabilisce sanzioni efficaci e che impone un vero e proprio contratto di responsabilità.

un piano di attrazione degli investimenti per facilitare chi da fuori viene dentro. Siamo consapevoli che delocalizzare, è vero, non significa internazionalizzare, ma noi dobbiamo sanzionare chi si delocalizza, ad esempio, dopo avere preso benefici, come è per la norma già vigente dal 2014, evitando quella specie di pubblicità legislativa che parla di sanzioni pecuniarie che duplichino o arrivino a quadruplicare il livello della sanzione economica a danno del beneficiario. Infatti, voi poi affidate il processo di recupero agli uffici periferici del MISE, che sono le camere di commercio e che non hanno, su questo, nessuna previsione finanziaria per reggere il contenzioso. Non vi potete aspettare che il sanzionato stia lì come san Pancrazio, che dice di sì davanti a ogni tentativo di recupero. C'è allora una norma che già sanziona, c'è una norma che prevede il periodo entro il quale va tenuto un comportamento virtuoso. Deve essere potenziato il lavoro che già è stato fatto in passato riguardante un piano di attrazione di investimenti

convenienze della pubblica amministrazione, implementando l'efficienza del sistema infrastrutturale; in una parola, si chiama contratto di sviluppo, che in Italia c'è, come strumento e istituto, ma dobbiamo fare sì che ci sia giacenza economica e finanziaria per dare ad esso ulteriore forza. Per questa ragione l'emendamento 05.2 punta a migliorare; potevamo anche solamente opporci, ma abbiamo voluto anche migliorare, scommettendo sul lavoro istruttorio delle Commissioni, che è risultato affannato, non adeguato e non all'altezza, perché avete impiegato soltanto alcune ore della vostra dedizione

trovi capienza e trovi sito. Per cui mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto di autonomia e di capacità istruttoria. Signor Presidente, l'intervento del senatore d'Alfonso, che ci richiama a temi molto alti, quale il rispetto della Costituzione e delle leggi, stimola una riflessione. Io vorrei chiederle, senatore D'Alfonso, se lei ha già ricevuto la lettera della Giunta per le elezioni e le immunità

queste cose non fanno bene alla reputazione della politica. Lei sa bene di essere incompatibile. Ha accettato di farsi eleggere al Senato...

e dei colleghi, soprattutto dei colleghi della Lega che con noi hanno condiviso un programma politico-elettorale di tutela del lavoro e dell'impresa, e per osservare che è certamente giusta la giusta lotta a chi agisce in base al principio del "prendi i soldi e scappa"

dettagliatamente gli errori contenuti nel provvedimento. Ieri il Vice Presidente del nostro partito, Antonio Tajani, ha quantificato in 130.000 i posti di lavoro

di questo decreto; altro che dignità! È il decreto miseria, bugia e disoccupazione! Votate i nostri emendamenti e buttate a mare un testo che fa del male all'Italia.

Seppure formulato in maniera ambigua, l'attuale comma 6-*bis* si presta a interpretazioni e di fatto conferisce una delega al Governo. L'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Ciò conformemente e in esecuzione del combinato disposto di cui agli articoli 76 e 77, La delega, quindi, può essere conferita soltanto mediante legge, mai tramite decreto-legge, che esproprierebbe il Parlamento della sua funzione principale, di cui all'articolo 70 della Costituzione.

chiedo al Governo almeno di poter trasformare in ordine del giorno l'emendamento 9.33 per avere una formulazione coerente con tutto il sistema in materia.

Presidente, l'intenzione con cui noi abbiamo lavorato anche nella legislatura precedente, a proposito di tutto quanto riguarda il gioco d'azzardo, non è mai stato solo ed esclusivamente orientato a una misura di tipo strettamente economico, ma sempre a tutela del giocatore fragile. Mi riferisco a quello che nella nuova dizione viene definito disturbo del gioco d'azzardo, che dovrebbe sostituire sia le parole «ludopatia» A me sembrava che anche l'istituzione del famoso numero verde, che è stato del tutto escluso e che mi auguravo si potesse trasformare in un ulteriore ordine del giorno, rientrasse nelle misure di tutela delle classi più deboli, che sono notoriamente, da un lato, gli adolescenti e, dall'altro, i pensionati. Intervenire su una funzione di questo tipo prendendosi in carica davvero i bisogni delle persone è più importante che non questa massiva e ossessiva attenzione, attenzione, che reputo auspicabile, ma impossibile da realizzare, sullo *stop* assoluto alla pubblicità perché, come in un altro emendamento sostenevo, ci saranno le vittorie straordinarie che riusciranno a incentivare la gente ad andare a giocare sempre e comunque. Tutte le misure di prevenzione richiedono un'attenzione molto forte, che è in capo più al Ministero della salute che non al Ministero del lavoro, a quello dello sviluppo economico o al MEF. Quindi, l'asse con cui noi abbiamo lavorato, anche spostando l'osservatorio

certamente è importante poter coinvolgere tutti quanti gli attori presenti sul territorio e tutte le articolazioni dello Stato impegnate a diverso titolo e con diversi compiti. Crediamo che questa battaglia, che si arricchisce di un ulteriore provvedimento, debba assolutamente coinvolgere le ASL e i servizi socio-sanitari territoriali. È per questo che, con l'emendamento 9-*bis*.1, chiediamo di poter inserire, all'interno degli spazi dedicati al gioco, una cartellonistica predisposta dalle ASL stesse, che evidenzi i rischi correlati al gioco d'azzardo. Chiediamo anche di segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza, tesi, da parte sia del settore pubblico che del privato sociale,

Chiediamo infine l'accesso degli operatori dei servizi dell'assistenza pubblica e del privato sociale negli spazi dedicati al gioco, perché, con la loro competenza e con le loro capacità, possano

al netto di tali considerazioni legate a questo specifico emendamento, mi preme sottolineare come il Governo, con questo provvedimento, abbia evidenziato che questi interventi legati al gioco d'azzardo siano delle prime misure, in attesa di un riordino complessivo del settore dei giochi. Qualcheduno in quest'Aula prima diceva che per le realtà complesse non si hanno soluzioni semplici. Ebbene, il rischio di queste pur positive misure è che, se noi le prendiamo singolarmente, le possiamo considerare...

direbbe un illustre collega - possono anche sembrare positive, ma il rischio è quello di una possibile inefficacia del loro insieme, perché, senza un'operazione che riguardi la possibilità di eliminare altre macchinette dalle sale gioco, queste misure legate alla pubblicità rischiano di essere assolutamente inefficaci. Voglio ricordare che i Governi precedenti sono riusciti a a portare da 378.000 a 265.000 le macchinette legate al gioco, con una riduzione superiore al 30 per cento. Certamente queste misure hanno un'efficacia importante, perché riducono gli spazi per il gioco. ben venga l'impegno, da parte del Governo, a operare in una maniera più completa su questo settore, ma vorrei ricordare al Ministro e Vice Presidente del Consiglio che a febbraio, durante la campagna elettorale, più volte egli si è espresso

che dichiarate di voler intervenire in maniera più organica su tutto il settore. Queste misure, che hanno una loro positività (lo ripeto), ma sono sganciate da provvedimenti tesi a ridurre in maniera significativa - come è già stato fatto nel recente passato gli spazi dedicati al gioco, rischiano di essere inefficaci. Vi chiedo quindi, nei provvedimenti che assumerete in futuro su questo tema, di considerare la gamma completa

Ovviamente ci auguriamo che siano ampliate e portate a livello nazionale, come anche il numero verde proposto dalla collega senatrice Binetti, sicuramente un'iniziativa

dilagare dell'azzardo sul territorio nazionale e l'aumento sconsiderato dell'offerta, che hanno portato avanti, in perfetta continuità, continuità, per vent'anni i Governi di centrodestra e di centrosinistra, hanno fatto diventare l'azzardo la seconda azienda italiana, con un milione di malati di azzardo e due milioni di persone a rischio. dire centrosinistra - molti dei quali avevano sottoscritto la proposta di legge per il divieto totale della pubblicità, nella scorsa Legislatura, senza vederla attuata, se non per quel ridicolo divieto parziale, che si è rivelato completamente inefficace. Abbiamo infatti visto il divieto della pubblicità, limitato alle televisioni generaliste e ad orari che addirittura non andavano neanche oltre la fine delle partite: quindi, se un ragazzino

i colleghi possano trovare difficile digerire che noi, dopo sessanta giorni, abbiamo già fatto quello che per anni hanno raccontato e non hanno mai concluso. Abbiamo affrontato delle *lobby*, che non hanno mai osato toccare e, anzi, le hanno assecondate per anni Governi di centrodestra e di centrosinistra, in perfetta continuità, come dicevo, dal cosiddetto decreto Abruzzo, che ha sdoganato le *videolottery*, facendo diventare gli abruzzesi i più più dipendenti dall'azzardo, invece che venire incontro ai danni del terremoto, al Governo Letta,

divieto della pubblicità, che era già nella delega fiscale ed è stato fatto saltare da un emendamento, approvato qui al Senato e proposto dal senatore Nencini; ci sono poi tanti altri esempi. Avete fatto qualcosina, qualche finta, come appunto il divieto parziale della pubblicità o la riduzione delle *slot machine*. È vero, avete iniziato la riduzione delle *slot*, ma, in sostanza, avete fatto quanto vi hanno detto ancora una volta i concessionari, ovvero spostare le offerte verso le *videolottery*, che sono molto più pericolose, e abbandonare un settore, che ha una filiera lunga e che ai concessionari rende poco, abbandonando così le *slot*, che non rendono. Se in un bar si passa da tre a due *slot*, semplicemente si concentra il raccolto nelle due *slot* che rimangono: non è quella la soluzione,

...iniziando ad invertire la tendenza, andando verso un calo costante dell'offerta e di conseguenza del raccolto, che riporterà il fenomeno ad un livello accettabile.

Presidente, io non capisco perché si voglia per forza polemizzare su un tema che dovrebbe vedere tutto il Parlamento consenziente nell'approvazione. Tra l'altro dagli interventi è emerso proprio questo, tranne la polemica fatta inutilmente dal ministro Di Maio quando disse che il centrosinistra era per le *lobby* del gioco d'azzardo. Con gli emendamenti presentati e con gli atti che abbiamo compiuto quando eravamo al Governo non avevamo nulla da dimostrare, ma siamo andati in una direzione totalmente opposta e mi meraviglia il fatto che la maggioranza non abbia votato queste proposte. L'unico elemento di contraddizione che noto è il provvedimento stesso che ci è stato presentato oggi. Ci dovete spiegare - lo chiedo soprattutto ai parlamentari di maggioranza intervenuti su questo tema come mai dite di essere contrari a questo tipo di intervento e favorevoli all'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo,

Dopo pretenderei un applauso anch'io, però.

Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il MAIE, movimento associativo espressione degli italiani nel mondo in questo Parlamento, apprezza e valorizza la volontà del Governo di dare un segnale che il Paese si sta veramente avviando verso un'epoca di riforme strutturali. Noi del MAIE riteniamo necessaria e benvenuta la semplificazione degli adempimenti in materia fiscale a carico di professionisti e imprese. In particolare, troviamo fondamentale l'iniziativa di combattere la precarizzazione del lavoro dei nostri giovani. Condividiamo anche la norma del decreto-legge rivolta a non permettere che le imprese percepiscano un aiuto statale e possano delocalizzare omettendone compromessi sociali e impositivi. Per ultimo, pensiamo che sia giusto abolire gli *spot* pubblicitari per il gioco d'azzardo: la ludopatia distrugge le famiglie e cause danni individuali e sociali gravissimi.

Signor Presidente, premetto che condivido gli obiettivi del decreto dignità che il ministro Di Maio ha riassunto in quattro punti: lotta al precariato, lotta alla ludopatia, lotta alle delocalizzazioni e alla sburocratizzazione. Quello che non mi convince è il vostro metodo. Non c'era l'urgenza per fare un decreto-legge, convocandosi in agosto e nel fine settimana, senza lasciare spazio alle opposizioni per apportare migliorie. Non mi convince neanche che, invece di cercare di migliorare tante cose che i vostri predecessori hanno fatto - come, ad esempio, il *jobs act*, che ha creato posti di lavoro - volete per forza cambiare tutto, perdendo quanto di buono ha fatto il precedente Governo. Temo che togliere flessibilità al mercato del lavoro distruggerà posti i lavoro, senza crearne di stabili. Il rischio di alimentare solamente il *turnover* e i contenziosi giudiziari è molto concreto. Inoltre, non ci convince la nuova normativa sui *voucher*, che è troppo stringente per il settore turistico e non sono state prese in considerazione le richieste del volontariato, del commercio, degli enti locali. Anche qui la fretta non ha permesso di scrivere una norma adeguata. Con un disegno di legge, ma anche con un approccio diverso nell'*iter* del provvedimento, noi crediamo si sarebbe potuta scrivere una legge all'altezza delle aspettative iniziali. Purtroppo così non è stato. Per tutte queste ragioni il nostro Gruppo esprimerà voto negativo.

non sosterremo il provvedimento in esame e voteremo contro, ma non per una ragione pregiudiziale; tutt'altro. Quando il ministro Di Maio, che in questo momento non vedo presente in Aula - probabilmente è in una pausa tecnica ha iniziato a delineare i contorni del decreto-legge, prima ancora di conoscerne il contenuto siamo stati incuriositi. La nostra curiosità è stata mossa dal lancio del decreto-legge, perché in quel lancio c'era un'ambizione molto forte, che noi condividiamo. Anzi, dico di più: dovrebbe essere un'ambizione condivisa da tutte le forze politiche in modo trasversale. L'ambizione era quella di immaginare uno strumento che fosse il primo passo, ma un passo importante, verso la lotta senza quartiere alla precarietà. E noi questo obiettivo lo condividevamo quando l'abbiamo ascoltato in questo Paese dovremmo iniziare a parlare di vero e proprio sfruttamento, in molti casi, in molte circostanze, in molti contesti. Così come erano sfruttati quei lavoratori che ieri hanno perso la vita nell'incidente che è stato ricordato anche in quest'Aula: è

e per il suo tramite ai membri della maggioranza e agli esponenti del Governo - c'è però una distanza molto forte, persino incolmabile, tra l'ambizione di quel titolo, la dignità, l'ambizione di quell'obiettivo e il contenuto di quel decreto-legge, gli effetti reali che esso dispiegherà. Intendiamoci: lo dico pensando che alcune misure contenute nel provvedimento vanno esattamente nella direzione che anche noi abbiamo auspicato in questi anni, un segnale di discontinuità rispetto a quelle politiche che non abbiamo condiviso - come, ad esempio, nella scorsa legislatura - quando incredibilmente un partito che avrebbe dovuto presidiare

- hanno rappresentato la prima vera, grande lacerazione tra quella proposta politica e un intero popolo. Parti di quel popolo poi hanno rivolto la loro attenzione - come è noto e come sappiamo - dal 4 marzo verso

Ed è una stretta giusta che vede il problema. Certo, se avessimo avuto una dialettica normale tra maggioranza e opposizioni e avessimo potuto esercitare la nostra funzione di parlamentari nella piena autonomia; ovvero se non avessimo incontrato quel muro che la maggioranza ha messo di fronte a una discussione che avrebbe dovuto essere più libera, forse qualche consiglio, qualche aggiustamento e qualche modifica sostanziale si potevano apportare anche a misure che hanno un

dei mesi, del tempo; per il fatto che la causa venga messa dopo i dodici mesi e non subito e l'aumento del contributo, si può innescare una sorta di meccanismo che, per effetto di eterogenesi dei fini, va esattamente nella direzione opposta a quella che si prefigge il Governo, e cioè anziché limitare l'uso e l'abuso del tempo determinato

La nostra banale previsione è che, non avendo messo mano a questo aspetto, nei prossimi mesi e nei prossimi anni si determinerà un aumento piuttosto drammatico dei licenziamenti per vizi di forma dietro i quali si nascondono evidentemente altri tipi di discriminazioni. Si trattava di accorgimenti che nessuno ha voluto prendere in considerazione, perché abbiamo fatto una discussione - come ho già avuto modo di sostenere ieri in un intervento - in Commissione nella nostra splendida solitudine di opposizioni e nell'assoluta afonia di una maggioranza passata dall'essere nella scorsa legislatura molto baldanzosa e, persino, a tratti rivoluzionaria ad essere ora connotata da *aplomb* istituzionale

Credo siano due gli aspetti esemplari rispetto alle questioni di cui forse avremmo dovuto discutere e dovremmo discutere nei prossimi mesi. noi siamo tra quelli che si sono opposti a una scelta molto scellerata e sciatta. Mi riferisco a quando l'ultimo Governo della scorsa legislatura ha cancellato con un tratto di penna i *voucher* perché aveva paura di essere investito da un *referendum* popolare promosso dalla più grande organizzazione sindacale di questo Paese. Ci siamo opposti perché bisognava fare un ragionamento più lucido e pacato. Bisognava - ad esempio - preservare l'utilizzo dei *voucher* per alcuni limitati ambiti di lavoro domestico, ma anche eradicare in modo definitivo quello strumento da tutti gli altri settori perché dall'agricoltura, alla ristorazione, ai servizi, al commercio il suo utilizzo ha rappresentato semplicemente un un meccanismo di moltiplicazione della precarietà e dello sfruttamento. E invece questo Governo ha pensato bene di mettere mano di nuovo a tale strumento, che tornerà drammaticamente a essere quello che è stato in passato: un moltiplicatore di abusi e di sfruttamento. C'è poi un poi un atteggiamento incomprensibile su questo punto, che non è tanto e solo determinato dalla distanza tra gli impegni che alcuni esponenti di questa maggioranza hanno assunto in passato ciò che invece non hanno fatto in questa circostanza. Mi riferisco in particolare all'impegno di ritornare a parlare nel nostro Paese della possibilità di reintrodurre l'articolo 18 sui licenziamenti illegittimi. È una scelta incomprensibile, perché penso che sarebbe stato un atto quasi dovuto tornare a parlare insieme, anche qui, trasversalmente alle forze politiche, della della possibilità che il Paese torni a essere un pochino più civile di quanto lascia oggi, in relazione alla necessità di introdurre uno strumento minimo di tutela, per cui un lavoratore, se viene licenziato senza giusta causa (e cioè illegittimamente), possa essere nelle condizioni di decidere lui stesso tra la monetizzazione del suo licenziamento

Ciò ha rappresentato un argine minimo per la civiltà giuridica del nostro Paese, e io dico per la sua civiltà. Non si è immaginato di ricominciare a parlare di questo tema, che non è un feticcio del passato, perché l'articolo 18 ha riguardato milioni di lavoratrici e di lavoratori. Averlo eliminato ha voluto dire non solo eliminare un diritto che spettava esattamente a quei lavoratori, ma anche aver ma anche aver reso più fragili i lavoratori che comunque non ne beneficiavano. I diritti nel mondo del lavoro sono un filo che lega le lavoratrici e i lavoratori e, se tu ne togli ad alcuni, anche gli altri diventano più deboli. Io penso che di questo bisognerebbe ricominciare a parlare. Lo dico - e chiudo davvero, signor Presidente - non perché penso che parlare di questo sia sufficiente per poter ricominciare a immaginare un futuro per il nostro Paese e la modalità con cui esso si risolleva. invece, che si debba chiudere la stagione nella quale si pensa e si è pensato, a destra e a sinistra, che, per far ripartire il Paese, occorra manomettere le regole del mercato del lavoro. No, torniamo a parlare di politiche industriali, di investimenti pubblici, di occupazione di qualità, di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Parliamo di tutto questo e, se lo facciamo insieme, credo che ridaremo sì dignità ai lavoratori, ma ridaremo dignità anche alla politica. Signor Presidente, premetto che siamo lieti di vederla al suo posto a presiedere quest'Assemblea.

il DNA di una forza di opposizione che vuole prima di tutto essere una forza di costruzione e proposizione. Quindi, se noi diremo "no" - come diremo - a questo decreto-legge, lo diremo motivandolo e soprattutto spiegando il perché. Al momento di tristezza che raggiungerà gli imprenditori non appena in queste ore verrà approvato il decreto-legge dignità, noi invece attireremo contestualmente delle proposte politiche concrete e a costo zero, che un'ora fa abbiamo presentato alla stampa con la nostra presidente Giorgia Meloni nelle aule parlamentari. Quindi, caro ministro Di Maio - che con piacere le vedo qui in Aula

un decreto-legge che, purtroppo - lo dico da cittadino prima che da politico - ritengo sarà il decreto della disoccupazione e del lavoro nero. Ho cercato davvero, senza pregiudizi, di calarmi nel vostro pensiero, nella lettura delle vostre norme e nella filosofia che le ha improntate e, al di là delle buone intenzioni che vi posso riconoscere, non sono stato davvero capace di intravedere un motivo

potrebbe essere stato da voi costruito in modo propedeutico ad un'altra filosofia, che non è quella di creare nuovi posti di lavoro e di creare fiato per le imprese e per la nostra economia, ma è quella piuttosto di arrivare alla decrescita felice. Se l'obiettivo è quello, allora forse ha

Altrimenti è difficile trovare dignità in norme che ragionano contro il mercato e contro le esigenze delle imprese, ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del nostro territorio e dalle quali, in queste ore - come sapete benissimo anche voi, cari colleghi - sta giungendo un grido di dolore, che arriva ad ogni senatore e ad ogni deputato. Non è tanto la Confindustria, che tante volte va a braccetto con la CGIL, come qualche volta avviene anche in queste Aule, ma sono le associazioni dei piccoli imprenditori che stanno rispondendo con rabbia a questa normativa restrittiva e sanzionatoria, a questi lacci e lacciuoli, che vengono apposti al mercato del lavoro.

Quindi, a prescindere dal merito, che tutti abbiamo evidenziato nei nostri emendamenti, anche la procedura tecnica di applicazione creerà problemi alle imprese. Quindi questa non è dignità, ma è un voler creare ostacoli a chi fa impresa. *voucher*, avete sì riaperto minimamente e blandamente a quei *voucher* che il Partito Democratico, sotto dettatura della CGIL, aveva eliminato,

di quelle che possono beneficiare dei *voucher*. Vorrei però chiedervi quante aziende alberghiere conoscete, a meno che non facciano ricorso al lavoro nero, che hanno fino ad otto dipendenti, perché già se ne hanno nove non potranno più ricorrere ai *voucher* nei picchi di lavoro e nei momenti di stagionalità. Non parliamo poi di quelle imprese che lavorano a fianco delle imprese alberghiere, come quelle della ristorazione e della pubblica somministrazione: tutte queste imprese sono escluse

Passando poi agli articoli successivi, parliamo della scuola. Qui avete una giustificazione: come bene ha detto il mio collega La Pietra questa mattina ci aveva già pensato la cosiddetta buona scuola

non dando risposta alle insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie, a tutte le sigle della categoria, che avranno inondato voi, come noi, con un altro grido di dolore, analogo a quello degli imprenditori, che citavo in

non si ostacola la delocalizzazione semplicemente aumentando le sanzioni; certamente si può fare anche quello, ma la delocalizzazione si ostacola soprattutto creando le condizioni perché l'imprenditore resti a produrre nella nostra Patria, in Italia, sia avvantaggiato nel produrre con i nostri prodotti,

Dobbiamo rispondere alla delocalizzazione premiando quegli imprenditori che producono in Italia, che usano materie prime e semilavorati per lo più italiani e che, soprattutto, facciano utilizzo di manodopera italiana. Così si fa per rispondere alla delocalizzazione; questo vuol dire essere propositivi e costruttivi. Passando agli articoli successivi, l'articolo 8, che cito brevemente, contiene delle altre restrizioni. Si tratta, quindi, di un decreto-legge fatto di restrizioni, lacci, vincoli, lacciuoli e restrizioni su ricerca e sviluppo. Non credo serva spendere parole e tempo per dire quanto fosse inopportuno restringere il credito d'imposta su ricerca e sviluppo.

in materia di giochi e di ludopatia siete stati bravi, avete rotto un muro di omertà, ve ne do atto. Mi auguro però che siate coerenti con quello che avete detto e scritto e che sappiate da oggi in poi, da qui all'autunno, dare veramente il la ad una stagione di chiarimento su questo tema, su questi interessi spesso occulti che si annidano verso chiunque cerchi di scoperchiare il sistema della ludopatia e dei giochi. Noi abbiamo nel nostro Gruppo il senatore il senatore Zaffini che in Umbria è stato abile estensore della legge contro la ludopatia, quindi siamo a disposizione. Abbiamo presentato in Senato un disegno di legge che vi invitiamo a calendarizzare e a discutere insieme a noi.

lo avete concesso a noi professionisti e non a quell'impresa che invece, in crisi di liquidità, aveva davvero bisogno della sua abolizione. Mi riferisco soprattutto a quelle piccole imprese in cronica

farà forse piacere a qualche sindacalista e a qualcuno che ancora ragiona nell'ottica veterocomunista degli anni Settanta; diciamo no ad un decreto-legge che, annullando il lavoro, sarà sicuramente propedeutico al reddito di cittadinanza; ad un decreto-legge che in sostanza si ispira al motto: meno impresa e più assistenzialismo. Tuttavia, poiché noi crediamo sempre nella buona fede di tutti, auspichiamo di vedervi nei prossimi mesi con delle variazioni al testo in discussione e con delle proposte che siano più vicine all'impresa, al lavoro e a tutti i cittadini.

rappresentanti del Governo, autorevoli colleghi, innanzitutto permettetemi di fare una segnalazione importante anche alla Presidenza, oltre che al Governo, sulla umiliazione che ha subito

il presupposto che tali provvedimenti possano essere discussi, analizzati e che vi possa essere un confronto serio e produttivo all'interno della Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Voi lo avete impedito, avete impedito la discussione! Per quale motivo, signor Ministro (perché l'ordine sarà arrivato sicuramente da lei)? Per non fare tardi stasera? Per anticipare di qualche ora le vacanze dei colleghi o per quale motivo? Probabilmente per non voler ascoltare le proposte di tutte le opposizioni. Questo è stato - mi permetta, signor Ministro - un grave errore da parte vostra e da parte di tutta la maggioranza. Io credo che l'atteggiamento che abbiamo dimostrato in Aula meritasse ben altro. Voi avete fatto peggio che mettere la fiducia, perché voi sì che avete messo il bavaglio alle opposizioni. PD)*. Mi permetta, signor Vice Presidente del Consiglio, mi deve togliere una curiosità: vorrei sapere qual è il nesso logico che accomuna un testo pasticciato, pieno di norme incongrue come il decreto-legge che stiamo votando, con il termine «dignità». Sfido chiunque a trovare, all'interno di questo testo complicato e farraginoso, qualcosa di degno: non c'è niente di degno. Siete stati ottimisti, ad esempio, nelle tabelle che voi stessi avete prospettato quando avete parlato di 80.000 posti di lavoro per difetto che il Paese avrebbe perso. Forse sono 100.000, alcuni colleghi delle altre forze di opposizione sostengono che saranno 130.000. È una cosa mai vista nella storia della Repubblica: si fa addirittura un decreto-legge, si chiede l'urgenza per far perdere posti di lavoro al nostro Paese e voi parlate di dignità? come sia possibile. Tra l'altro lo hanno spiegato molto bene - credo - le associazioni imprenditoriali di tutto il Nord produttivo, una terra che dovrebbe interessare particolarmente a una forza importante della maggioranza, la Lega. Imbastiamo anche contro di loro, contro i rappresentanti di questa associazione delle imprese e degli imprenditori una bella macchina del fango *social* come quella che avete organizzato contro il professor Burioni sui vaccini? È questo il modo in cui si fa politica? Io credo che gli imprenditori meritino di essere ascoltati. Dopo l'approvazione di questo provvedimento, succederanno due cose: la prima è che aumenterà il *turnover*, per non rischiare il contenzioso con il ripristino che voi avete voluto delle causali;

Voi non lo potete chiamare decreto dignità, perché questo è proprio il decreto della disoccupazione, così andrebbe chiamato. era diversa, magari più complessa e anche più difficile da comprendere, da trasmettere e da comunicare ai nostri concittadini. Parlava di scuola-lavoro, di un percorso formativo che preparasse in maniera adeguata anche all'ingresso nel mondo del lavoro; parlava di incentivi all'investimento per le imprese, in particolare agli investimenti tecnologici e basati sull'innovazione, parlava di agevolazioni per il lavoro a tempo indeterminato; parlava di garanzie crescenti per il lavoro e per i lavoratori. Avete messo in piedi, invece, un meccanismo infernale che rischia di legare le mani alle imprese, con la conseguenza ovvia di aumentare la disoccupazione e il ricorso al lavoro nero: questo avete fatto. Dovevate concentrarvi sulla questione centrale della competitività del Paese, con politiche industriali serie e condivise. Vede, signor Ministro, lei poteva venire in Aula a proporre al Paese una diminuzione del cuneo fiscale, poteva proporre il salario minimo, poteva proporre una buonuscita per i lavoratori che venivano licenziati dopo il tempo determinato, gli incentivi alla stabilizzazione

non di aumentare le tasse alle imprese, di aumentare la burocrazia, di aumentare le causali, di aumentare il contenzioso, di aumentare la precarietà e di aumentare, ripeto, il lavoro nero. *(Applausi dal Gruppo non di una discussione inutile e totalmente ininfluente sul mercato del lavoro italiano. Invece questo provvedimento vuole mettere in contrapposizione il lavoro e l'impresa, facendo un danno al lavoratore e un danno alle aziende. PD)*. Con quale coraggio si parla di dignità, lo ripeto, per un provvedimento che casomai toglie, perché riduce i posti di lavoro? Ma lei, signor Ministro, mi permetta, conosce il lavoro? Conosce l'impresa, le imprese? Lei ha provato la soddisfazione di essere assunto la prima volta, la soddisfazione della prima busta paga, della conferma a tempo indeterminato? Lei sa di cosa si parla, signor Ministro? Per favore, fate terminare il senatore Marcucci.

Ecco come combattete la precarietà, signor Ministro: aumentando i licenziamenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Diciamoci la verità. Questo Governo aveva un solo obiettivo, in particolare per voi del MoVimento 5 Stelle: questo unico obiettivo era un argomento per andare sui *social* e sui telegiornali,

Vogliamo parlare velocemente degli altri effetti che questo decreto-legge produrrà. Avevate promesso di risolvere il problema delle maestre e dei maestri: *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avevate promesso di assumere i giovani e li escludete, propri i giovani laureati in scienze della formazione primaria, dal vostro concorso straordinario. Noi vi abbiamo proposto una soluzione per garantire la continuità didattica, quella vera, e ne avete fatto carta straccia. Ci dite di voler potenziare i nidi e la scuola dell'infanzia e invece non volete aumentare gli organici. E poi, sul gioco d'azzardo, signor Ministro e signor Presidente del Consiglio, a parole fate retromarcia per combatterlo, ma poi vi rivelate per quello che siete, con le vostre vere intenzioni, e aumentate le previsioni delle entrate finanziarie, aumentate le tasse sul gioco: vi volete finanziare con il gioco d'azzardo, questa è la verità. Lo ripeto, purtroppo, signor Presidente del Consiglio e signori Ministri, ci stiamo abituando a questo tipo di politica, a questo vostro modo di far politica. State cercando di bloccare la RAI da settimane per una poltrona in più, fregandovene della pluralità dell'informazione e dei diritti del Parlamento. Siete venuti con i vostri Ministri in Aula, in particolare con il ministro Salvini e il ministro Bonafede, che è presente anche oggi, ad offendere il Parlamento. Tanto vale l'auspicio del vostro *leader* Casaleggio, che lo vuole chiudere. State bloccando un imponente piano di investimenti, fatto per modernizzare il Paese (certo, la TAP, la TAV, ma anche molte altre opere infrastrutturali), che avrebbero potuto cambiare l'Italia, avrebbero potuto modernizzarla. Avete chiuso la

Signor Presidente, signor Primo Ministro, signori Ministri, gentili colleghi, sono grato al Capogruppo che mi ha dato la possibilità di svolgere un intervento politico dopo tre giorni di lavoro istituzionale. Preciso che è stato per me un onore e mai un onere presiedere le Commissioni congiunte 6a e 11a. Che il comportamento dell'opposizione sia stato ostruzionistico lo hanno ammesso, con franchezza e lealtà, gli stessi colleghi, come risulta fedelmente dai resoconti sommari di seduta e com'era ampiamente loro diritto fare. Ma si è trattato di un ostruzionismo civile, rispettoso del Regolamento e - permettetemi di dirlo - in alcuni casi anche spiritoso nei modi, cosa che ho particolarmente apprezzato, soprattutto nel collega Mauro Laus cui vanno i miei auguri di buon compleanno. In questo contesto non facile ho cercato di rendere costruttivo questo ostruzionismo, mantenendo la calma e riconoscendo le ragioni dell'avversario, cosa un po' inattesa in quel pericoloso *skinhead* del quale vi racconta oggi la stampa. L'urgenza del provvedimento c'era e c'erano anche i numeri per sostenerla, come hanno dimostrato le votazioni. Ho dichiarato in Commissione - e lo ripeto qui - di capire, e in parte anche di condividere, la frustrazione di chi avrebbe voluto sinceramente contribuire a migliorare un testo scritto da uomini e quindi per definizione perfettibile. Dichiaro solo qui e senza polemica che questa legittima aspirazione mi sembra però logicamente incompatibile con il fatto di aver presentato oltre 700 emendamenti dopo aver votato un certo calendario d'Aula e dopo essersi accordati su un orario di deposito emendamenti

Non voglio essere polemico. Desidero solo sottolineare il valore pedagogico delle sconfitte in democrazia. Del resto, anche per me, aver portato il testo in Aula senza relatore non è esattamente una vittoria, dopo tanti sforzi di mediazione e di ascolto, ma va bene così. Forse dalle sconfitte qualcosa si impara: sono passati 611 giorni dal 4 dicembre 2016 e il PD valorizza il bicameralismo. Confido che intorno al 5 novembre 2019, a 611 giorni dalla sconfitta del 4 marzo scorso, il PD possa trarne le giuste conseguenze e capire che non ha perso perché gli italiani sono razzisti per colpa di Salvini e assumere, anche in Assemblea e nel Paese, quei toni propositivi e costruttivi che finora gli ho visto e gli riconosco con estrema gratitudine solo in Commissione. Voglio dire con grande chiarezza che chi dipinge l'Italia del 2018 come fosse l'Alabama degli anni Cinquanta non facilita il nostro lavoro, non rende un favore al Paese e neanche a se stesso. Infatti, poi fallisce. Quindi, fatto salvo il rispetto per tutti i lavoratori, giornalisti inclusi, e il loro diritto a una retribuzione che garantisca loro un'esistenza libera e dignitosa, voglio dire al corteo delle ipocrite prefiche del pluralismo, che si ha pluralismo quando l'informazione veicola una pluralità di opinioni diverse, come ho cercato di fare io nel mio piccolo e come fa l'illustre Presidenza di questa Assemblea, non quando una pluralità di mezzi viene dispiegata per veicolare un'unica opinione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Quella opinione che noi, con una certa sopravvalutazione pomposamente chiamiamo pensiero: il pensiero unico. E qual è questo pensiero unico? È la religione di quello che il vice *premier* Di Maio ieri ha chiamato il dio mercato. Su questi temi mi piacerebbe e mi piacerà, in un clima svelenito, confrontarmi con i colleghi del PD e dell'opposizione in generale, perché la religione del mercato chiede atti di fede, ma propone dogmi incoerenti. Nella discussione di questo decreto-legge le nostre opposizioni ci hanno imputato diverse volte un atteggiamento punitivo verso le imprese, ma ho sentito queste stesse opposizioni elogiare tante volte il progetto di moneta unica, perché alzando l'asticella del cambio avrebbe spronato le imprese a essere più competitive. E questo non è forse un atteggiamento punitivo, una specie di darwinismo economico per cui si salva chi può e gli altri imprenditori, soprattutto se sono piccoli, devono scomparire perché inetti a vivere? *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e se la rigidità del cambio ha questa funzione pedagogica, perché non dovrebbe averla anche la tutela e quindi una ragionevole rigidità del salario? In un'economia di mercato è il prezzo a segnalare il valore delle risorse: capitale e lavoro. Svilire il lavoro umano con remunerazioni indecenti porta necessariamente con sé un calo della produttività, da due lati: quello del lavoratore, perché, ci come ha insegnato Stiglitz, un salario decente incentiva il lavoratore; quello dell'impresa, perché un costo troppo basso non incentiva un uso più efficiente delle risorse. Tanti studiosi hanno approfondito questa tematica. In proposito, desidero citare, in particolare, il collega amico Pasquale Tridico. Confindustria - ci dicono - non è contenta.

dimostra grande generosità (non lo vedo in Aula e lo saluto, è stata una piacevole conoscenza). Dico questo per capire l'autorevolezza delle previsioni. Per aiutarci a elaborare il lutto di questa augusta disapprovazione, fatemi fare qualche nome: Fiat, Sky, Luxottica, Marcegaglia, Honda Italia. Cosa sono? Sono alcune delle grandi aziende che ultimamente hanno abbandonato Confindustria, un'associazione che ormai rappresenta solo il mondo della grande impresa (e di una certa grande impresa) e al cui interno hanno molto peso le grandi partecipate pubbliche, che sono certamente delle imprese vitali e strategiche in un'ottica di sistema, ma sono pur sempre lontanissime dalla piccola e media impresa che costituisce il nucleo del nostro sistema imprenditoriale. *(Applausi dai noi ci chiedono di favorire la flessibilità in uscita dei lavoratori, ma di far aumentare la domanda interna, sburocratizzare la pubblica amministrazione e semplificare gli adempimenti fiscali. E bene ha fatto ieri il vice *premier* Di Maio a ricordare che le tutele dei lavoratori sono uno strumento per rianimare la domanda, perché rinsaldano la fiducia

tutte le voci, ma, colleghi, lasciate che attiri la vostra attenzione su un piccolo dettaglio, estraneo per merito, ma non per metodo. Le stesse associazioni e aziende che nella seconda metà di giugno, con un certo sprezzo verso l'interlocuzione già avviata con le forze di maggioranza, compravano pagine di giornali per esortare questo Governo a non toccare la legge 8 aprile 2016, la riforma delle banche di credito cooperativo), dopo l'approvazione del decreto milleproroghe si sono sperticate in complimenti per l'azione del Governo. Insomma, il Governo Conte è riuscito in un'impresa impossibile: migliorare una riforma,

Le nostre opposizioni in Commissione, in Assemblea e ovunque ci rimproverano di fare propaganda. Oggi il senatore Nannicini, che saluto e che ho imparato a conoscere e apprezzare nel lavoro di Commissione, con grande lucidità ha ammesso che la propaganda, come del resto l'ostruzionismo, è un dato fisiologico

non c'è alcuna necessità di limitare l'utilizzo contrattuale rispetto ad altre in quanto la precarizzazione in questo Paese non è causata - e non era causata - dall'impiego di alcune forme contrattuali rispetto ad altre, ma dal perdurare di una crisi economica che ormai si trascina da dieci anni. Quindi, le stesse premesse sono smentite dai numeri. Cifre che non fotografano, e non fotografavano, alcuna emergenza sul lavoro a termine e, quindi, alcuna impellenza (motivazione di decreto-legge) decreto-legge) di correre dietro a un testo che è rimasto sostanzialmente immodificato rispetto al testo proposto dal Governo,

che si riapre un conflitto storico tra capitale e lavoro. Parte del dotto intervento che mi ha preceduto richiama a tutto ciò. Lascio a chi lo vorrà di approfondire questa parte. Noi, come forza politica responsabile, abbiamo ascoltato le parti sociali, con giudizi molto negativi, da parte di tutte le parti sociali, anche di quelle parti sociali che non rappresentano la grande impresa o solo la grande impresa. Ad una disciplina complessa, che coinvolge gli interessi dei lavoratori e delle imprese, si è risposto con norme improvvisate che non necessitavano di alcuna urgenza. I numeri che ci ha presentato la relazione tecnica iniziale, che prospettava la perdita di ottomila contratti di lavoro, sono certamente stimati per difetto. E nonostante questo, e forse è la prima volta abbiamo assistito a ciò, la relazione è stata fatta da un ente che dipende direttamente dal Ministro proponente il decreto-legge. Di una cosa siamo sicuri. Al di là delle stime, la sola disincentivazione del lavoro a tempo determinato, attraverso i meccanismi di penalizzazione che abbiamo letto,

Certamente questa sarà una valutazione sulla legge di bilancio. Non entro adesso nel merito del 3 per cento e del rapporto con l'Unione europea. È una partita che, peraltro, ci vede

(che alla Camera lo stesso Governo ha prorogato), molte aziende hanno scelto il contratto a tempo determinato, perché era la tipologia contrattuale che più si confaceva alle prospettive di crescita di quelle imprese,

ufficiali, che vedono oggi l'attivazione di 60.000 contratti a tempo indeterminato, grazie ai 162 milioni di incentivi ora introdotti, non ci dicono quanti se ne sarebbero attivati ugualmente senza incentivi. Così non funziona e non possiamo partire dal concetto di condannare le piccole e piccolissime imprese, quelle dell'artigianato, del commercio e della manifattura, che non sono rappresentate da Confindustria, collega Bagnai,

vieta ai contratti a tempo determinato di diventare poi a tempo indeterminato. Subire però penalizzazioni perché si dà lavoro è l'ultima cosa che chiedono gli imprenditori, così come perdere il lavoro.

per regolarizzare il più possibile lavori che non hanno la possibilità di continuità e che ben vanno incontro - anche per i soggetti pubblici, se saranno introdotti - aiutare le fasce più deboli. Non su tutto; alcuni sono stati posti, a livello molto limitato, purtroppo, per poche categorie, creando peraltro discriminazioni tra soggetti similari. Credo sia dimostrato che ricorrere solo alla regolamentazione delle forme contrattuali non risolve il problema. È l'economia che cresce che crea il lavoro, è la fiducia degli imprenditori,

Al contrario, ritenevamo un'occasione utilizzare il decreto-legge per risolvere la questione scuola, per dare percorsi di certezza ai docenti anche delle scuole paritarie.

hanno delocalizzato dopo aver percepito gli incentivi, si rischia di minare il processo di internazionalizzazione del nostro Paese, delle nostre imprese e delle più piccole imprese.

forse anche 130.000, come citavano gli ultimi dati - che non si vedranno più rinnovato il contratto di lavoro. Per questi motivi, noi votiamo contro.

membri del Governo, presidente Conte, illustri colleghi, nell'ampio dibattito parlamentare che si è svolto su questo decreto-legge, in Assemblea e nelle ventisei ore di Commissione, ci sono stati diversi spunti di vero interesse che questa maggioranza ha ascoltato, ma sono anche state usate parole che faccio difficoltà a collocare in questo dibattito. Si è parlato di decreto indignità e di vergogna:

Dovremmo vergognarci di aver posto un ulteriore freno a imprese che vengono a sfruttare i lavoratori e gli aiuti su questo territorio per poi delocalizzare e lasciare in strada le persone? Io credo di no, non dovremmo vergognarci. *(Applausi

del gratta e vinci? Credo che non dobbiamo vergognarci di aver tolto questa umiliazione a quella famiglia. Credo che dobbiamo esserne orgogliosi. Colleghi, questo provvedimento non esaurisce i temi che tocca, ma porta al centro un'alta dimensione politica perché aggredisce i problemi,

Penso ad Angelo, che faceva il magazziniere in una grande multinazionale, che una mattina è andato a beggiare e non ha trovato più il *badge* funzionante, perché quella multinazionale adesso produce a otto fusi orari da questo Paese. Penso a Marisa, che ha un figlio che è sul un figlio che è sul baratro per colpa del gioco d'azzardo. Su questo tema oggi abbiamo messo al centro alcuni dei problemi che ci sono, grazie anche al lavoro che è stato fatto nella precedente legislatura da alcuni colleghi: penso a Giovanni Endrizzi e a Matteo Mantero, che sono qui e che hanno lavorato con la Caritas e con le associazioni su questo problema. Dicevo, abbiamo aggredito dei temi. Penso a chi, ad esempio, ha una partita IVA. Io ripenso a quando, vent'anni fa, mio padre, che faceva il commercialista, spariva il 1° maggio e rientrava il 31 maggio: era quello il momento in cui i commercialisti concentravano degli adempimenti, come il famoso 740. Penso

ministro Di Maio, io la ringrazio, perché è stato qui ad ascoltare il dibattito parlamentare, cosa che non credo sia una consuetudine in queste Aule. Ma la ringrazio anche perché ci dà la possibilità, aggredendo questi temi, di tornare sui nostri territori, poter guardare negli occhi queste persone e dire che oggi c'è qualcuno che si occupa dei loro problemi. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Finalmente Paolo, Angela, Marisa non avranno più un riferimento lontano che non percepiscono, ma un Governo che cerca di interpretare i loro problemi e di risolverli attraverso i provvedimenti, che è quello che dovrebbe fare la politica sempre. Io ritengo che il dibattito si sia concentrato anche un po' troppo sulla questione dei posti di lavoro in meno o in più. quando mai un provvedimento giuslavorista incide sulla creazione dei posti di lavoro? È un provvedimento che tratta dei diritti dei lavoratori: è soltanto questo il tema. Il diritto del lavoro è il tema che si tratta con questi provvedimenti. Quando parleremo di sviluppo economico e delle idee che questo Governo ha in proposito, è allora che andremo a porre le condizioni per creare nuovi posti di lavoro. Ma non era certo questa l'intenzione odierna: oggi volevamo rimettere al centro i diritti dei lavoratori. Perché noi riteniamo che bisogna invertire la rotta e far sì che, siccome la mia generazione sta peggio di quella precedente, i nostri figli invece abbiano un'idea di futuro e una prospettiva migliore di quella di oggi. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato elemento di coesione sociale in questo Paese. M5S)*, perché garantiva la possibilità di farsi un mutuo, la possibilità di farsi una famiglia, la possibilità di fare una spesa, la possibilità di andare in vacanza. Io penso che l'ossatura economica del Paese non siano le grandi imprese. Noi abbiamo una piccola, micro e mini impresa, lavoratori e artigiani che hanno

e anche, se mi consente, assaporando questo gusto per la seconda volta in meno di due mesi di approvare una conversione in legge senza ricorso alla fiducia, che dichiaro con grande onore il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. Grazie

È uno spettacolo al quale non vorrei mai assistere. Togliete i cartelli. Non siamo all'asilo.

e diversa. Non siamo all'asilo con i cartelli. Non stiamo giocando. Siamo nel Parlamento dove ognuno esprime ciò che vuole, per grazia di Dio.

Senatori colleghi, in questo inizio di legislatura l'Aula del Senato ha avuto modo di ricordare e onorare la memoria di autentici eroi civili della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, magistrati che per questa causa, insieme alle donne e agli uomini della loro scorta, hanno pagato un tributo altissimo, che non si sono mai piegati, che sono stati esempio di rettitudine e di alto senso dello Stato, ai quali l'Italia di ieri e di oggi deve molto. Uomini come Antonino Scopelliti, magistrato chiave nella lotta alla mafia e uno dei più apprezzati procuratore di Cassazione, che il 9 agosto del 1991

da quel tragico giorno siamo ancora lontani dal vedere scritta una parola definitiva di verità sull'omicidio Scopelliti. Di certo c'è solo che venne ucciso perché era temuto, perché scandagliava, approfondiva, perché aveva un forte senso della giustizia e della legalità. In altre parole, faceva il suo lavoro. Grazie alla fondazione a lui intitolata, ogni anno la memoria di Antonino Scopelliti viene rinnovata attraverso il ricordo delle sue azioni perché quella cultura della legalità per la quale si era sempre battuto possa definitivamente attecchire tra le nuove generazioni e soprattutto tra i giovani di una terra martoriata, dove il germe della criminalità organizzata è ancora vivo, come la Calabria. Invito tutti a un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, colleghi senatori, permettetemi subito di dire che il Governo in queste ore è vicino alle famiglie delle vittime e dei feriti, sia moralmente che fisicamente. Lo prova la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi, sia a Bologna che a Foggia. Non è concepibile dover assistere a scene sconvolgenti come quella che abbiamo visto e rivisto ieri. Non è accettabile. Permettetemi una parentesi anche sull'incidente in Puglia: si è ripetuta, in termini ancora più gravi, una tragedia che è un film già visto, dopo lo scontro stradale di sabato scorso. Quello di ieri, prima di essere un gravissimo incidente, è il capitolo estremo di una storia orribile di sfruttamento, una forma moderna di schiavitù che in questo Paese non possiamo tollerare. Il caporalato va debellato e ha fatto bene il ministro del lavoro Luigi Di Maio a riferirsi a un'intensificazione dei controlli contro il lavoro nero, attraverso un maggior numero di ispettori. È assurdo che serva una tragedia per mettere sotto i riflettori un fenomeno che, anno dopo anno, stagione dopo stagione, raccolta dopo raccolta, offende quel senso di umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi. Quei sedici ragazzi erano venuti in Italia per avere un futuro migliore e invece hanno trovato la morte. I dodici deceduti ieri viaggiavano probabilmente in piedi e stipati, complessivamente in quattordici, dentro un furgoncino che poteva portare al massimo otto persone. Tornando sui fatti di Bologna, ieri, 6 agosto, alle ore 13,50, il comando dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata per l'esplosione di una autocisterna da 25 metri cubi sull'autostrada A14, all'altezza di Borgo Panigale (Bologna), sul cavalcavia

alla guida del tir della ditta Loro Fratelli di Lonigo, in provincia di Vicenza, che ha tamponato il camion poi esploso e ha causato circa 145 feriti. Numerose le vetture incendiate, che per la maggior parte appartengono a due autoconcessionarie vicine. I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio che è divampato dopo lo scontro. Una volta spente le fiamme, è stato necessario raffreddare l'area e continuare la ricerca e la localizzazione di altre vittime o feriti. I feriti sono stati immediatamente trasportati nelle strutture ospedaliere più vicine. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato dal conducente della ditta del mezzo che trasportava GPL. Il carico ha preso fuoco e ha dato il via a una serie di esplosioni a catena, che hanno interessato la vicina caserma dei Carabinieri di Borgo Panigale, determinando il ferimento di undici carabinieri. Sono altresì rimasti feriti tre poliziotti. Grande merito va alle Forze dell'ordine, per aver evitato conseguenze peggiori con il loro pronto intervento. *(Applausi)*. Dalle immagini registrate dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, il camion sembrerebbe non aver frenato, nonostante la coda segnalata, finendo su un mezzo fermo che trasportava fusti di solvente. Il conducente di questo tir, rimasto ferito, si chiama Antonio Verdicchio di San Felice a Cancello, nato nel 1973. Il tamponamento ha coinvolto anche una bisarca, il cui conducente, ferito anch'egli, di nazionalità rumena, classe 1976, si chiama Silviu Partenie. Il tamponamento ha innescato l'incendio che, dopo circa quattro minuti, ha provocato l'esplosione della cisterna, che a sua volta ha determinato il crollo della sottostante infrastruttura. Nel corso della notte sono state effettuate, da parte della società Autostrade per l'Italia, tutte le verifiche tecniche, corredate di prove di carico delle infrastrutture adiacenti, che hanno dato esito favorevole e che non hanno evidenziato nessun tipo di problema sulle parti strutturali della medesima opera adiacente le parti crollate. Pertanto, nella notte è stato possibile ripristinare la pavimentazione danneggiata della carreggiata nord dell'autostrada adiacente a quella dell'incidente e predisporre la segnaletica e le delimitazioni di sicurezza per la riapertura dell'autostrada, che è avvenuta stamattina alle ore 9,10, a corsia singola in scambio di carreggiata. Contestualmente è stata riaperta anche la tangenziale in direzione Casalecchio. Al momento resta quindi chiusa esclusivamente la tangenziale in direzione opposta, limitatamente al tratto compreso tra lo svincolo 2 e lo svincolo 3. Ciò costituisce una prima risposta importante, anche se parziale, dopo la tragedia, al fine di rendere più fluido il traffico, considerato l'esodo estivo. In merito all'intervento di ricostruzione, Autostrade per l'Italia sta verificando presso i principali produttori nazionali ed europei la disponibilità in pronta consegna di 12 travi con interasse appoggi di 24,65 metri e con altezza di 1,10 metri. Tale eventuale disponibilità consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi della ricostruzione, altrimenti stimabili in non meno di cinque mesi. Circa i costi di ripristino dell'esistente, la società Autostrade per l'Italia informa che, al momento, sono quantificabili in via di massima in un milione di euro, comprensivi degli interventi di demolizione e provvisionali. Le simulazioni sul traffico ci dicono che con l'attuale situazione non avremo disagi in autostrada fino a settembre. Siamo sicuramente di fronte ad una grande tragedia, che ha coinvolto non solo un tratto autostradale, ma un intero quartiere della città di Bologna. Come Governo stiamo monitorando minuto per minuto la situazione e stiamo cercando di ripristinare livelli sufficienti di circolazione. Esperti del mio Ministero, unitamente a tre Sottosegretari di Stato, sono sul luogo dell'incidente. La nostra presenza lì vuole essere un segno di vicinanza mio e di tutto il Ministero a fianco dei familiari delle vittime e dei feriti. Continueremo ad essere presenti sul luogo dell'incidente per seguire da vicino gli sviluppi della vicenda e fare luce su questa ennesima tragedia. Forze dell'ordine, Forze di polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco, Prefettura, Comune e Ministeri, ciascuno attraverso gli uffici competenti, sono al lavoro in coordinamento tra di loro per fare tutto ciò che è necessario. Poche ore fa si è tenuto un *summit* operativo in Prefettura, anche per individuare la disponibilità dei siti per poter procedere alle operazioni di demolizione delle parti instabili dell'infrastruttura e alla rimozione di materiali franati sulla sottostante via Bragaglia, operazioni propedeutiche all'intervento di ricostruzione della sede autostradale. Intanto, ho già espresso la mia ferma volontà di agire su due fronti. Da una parte, vi è la necessità di alleggerire il traffico merci su gomma e, in aggiunta, la necessità di dotare i tir di tecnologie che riducano al minimo la possibilità di errore umano. Questo Ministero vuole quindi incentivare l'installazione sui mezzi che trasportano merci pericolose - che superano le 35.000 unità, secondo i dati in nostro possesso - di presidi di guida assistita. Sto parlando di dispositivi anticollisione, frenata automatica, controllo predittivo della velocità, ritrovati ormai abbastanza comuni nelle nostre auto più nuove e che non possono non corredare questi mezzi pesanti, che rischiano ogni momento di trasformarsi in ordigni ambulanti. Al riguardo, il mio Ministero sta dando un forte *input* alla sperimentazione su strada delle soluzioni di *smart road* e di guida connessa ed automatica e sta introducendo, tra l'altro, sistemi di interazione tra veicoli e infrastrutture, capaci di veicolare informazioni e servizi di interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida guida e del traffico, nonché sistemi per l'interazione e la collaborazione tra veicoli. Occorre assicurare massimi *standard* di sicurezza; esistono già norme specifiche abbastanza aggiornate, riguardanti il trasporto su strada di merci pericolose, anche profilate in base alla tipologia di materiale. Verificherò comunque se le regole siano state rispettate. Inoltre, il mio Ministero e il Governo lavoreranno in sede di discussione europea sul pacchetto mobilità, affinché si trovi un giusto equilibrio tra le condizioni di lavoro dei conducenti e la libertà di prestare servizi transfrontalieri per i trasportatori. Bisogna contemplare una corretta ed equa alternanza tra tempi di guida e tempi di riposo, assicurando piena tutela ai lavoratori della strada. tutela è troppo spesso messa in discussione da forme di concorrenza sleale, che penalizzano le nostre imprese dell'autotrasporto. Infine, vorrei sottolineare che non consento a nessuno di strumentalizzare in modo becero e vergognoso quanto accaduto ieri a Borgo Panigale collegando indebitamente l'evento luttuoso al dibattito circa determinate soluzioni infrastrutturali, che riguardano l'area bolognese. Si tratta di un *dossier* su cui questo Ministero sta lavorando duramente, allo scopo di garantire anche in

Signor Presidente, ridurrò al minimo le considerazioni perché in cinque minuti non si può dire molto. Innanzitutto apprezzo il fatto che questa mattina il Presidente del Consiglio sia andato a Foggia e a Bologna,

Io credo che in quest'Aula condividiamo tutti le sue parole. Su questo non ci si può dividere: vedere persone, esseri umani, con la loro dignità, ammassati su un camion di questo tipo

io purtroppo ho sentito altre volte parlare di questo e mi auguro che si possa fare veramente più controllo e più prevenzione. Vorrei dire una cosa a tutti i colleghi: noi spesso vediamo il fenomeno degli extracomunitari clandestini che sono nel nostro Paese e lo biasimiamo, al di là delle posizioni politiche che si hanno in quest'Aula. Bene, non dimentichiamoci mai - e questi fatti ce lo riportano duramente - che dietro a tanta clandestinità,

non possiamo fare una valutazione serena e seria su tutta la vicenda. Quella accaduta a Bologna è, per ovvie ragioni, la vicenda che mi ha portato ieri a prendere la parola in quest'Aula dopo le prime notizie. Credo sia giusto rivedere le normative sui carichi pericolosi ed è bene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti metta in atto dispositivi per sperimentare nuovi meccanismi di sicurezza. Non sono un esperto, ma certamente è tutto positivo. È bene anche che ci sia stata una risposta tempestiva e immediata per ripristinare viabilità e demolire ciò che va demolito. Non dimentichiamo, colleghi, che un quartiere di Bologna è stato semidevastato. quindi, un problema di indennizzo immediato per i familiari delle vittime; c'è un problema di cittadini coinvolti nelle loro abitazioni, con case che hanno subito gravi danni o che sono parzialmente inagibili; c'è un problema di aziende e realtà produttive che sono state devastate da questa esplosione e che pertanto vanno risarcite. Io credo che il Comune di Bologna, la Regione e lo Stato non siano tre realtà isolate realtà isolate l'una dall'altra; sono tre realtà chiamate, in questo caso, a esercitare una leale collaborazione tra poteri dello Stato per dare una risposta, in termini di risarcimenti ed indennizzi, che deve essere il più possibile rapida, perché non si possono tollerare i tempi che purtroppo tante volte vediamo in vicende di questo tipo. Io non ho altro da aggiungere, salvo rivolgere un ringraziamento alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri e alla Polizia, che hanno di mostrato ancora una volta quanto importanti siano e con quanto spirito di abnegazione difendano i cittadini. Un'ultima parola però me l'ha tirata lei, signor strumentalizzare in modo becero una vicenda di questo tipo per introdurre surrettiziamente una valutazione sul passante di mezzo sarebbe vergognoso. Credo che nessuno possa pensare realisticamente di utilizzare questa vicenda per porre una questione su cui noi - bolognesi, noi enti locali bolognesi, noi Regione Emilia-Romagna - stiamo cercando di interloquire con lei. però sa che il problema esiste. Io ho visto questo Governo atteggiarsi con molta coerenza. Ho sentito il Presidente della Regione Veneto e il Presidente della Regione Lombardia

sereno - che lo stesso metro venga applicato dal Governo per la Regione Emilia-Romagna, perché non ci sono parenti di serie A e di serie B, le Regioni sono tutte uguali, in un rapporto di collaborazione e di lealtà con il Governo centrale.

Per brevità, sottolineo l'affermazione che ha fatto il senatore Casini: è chiaro che qui ci sono gravi responsabilità di italiani, su cui bisogna intervenire. Il ministro Centinaio ci ha assicurato, proprio in seguito ad una nostra richiesta, che non intende modificare la legge sul caporalato,

Le cose che lei ha detto sono importanti, tenendo conto che siamo di fronte a un nodo strategico della viabilità. Va benissimo farsi carico di tutti i danni e lavorare per le nuove tecnologie, ma secondo me occorre anche pensare a nuove norme per quello che riguarda i trasporti pericolosi. benissimo usare le nuove tecnologie per la sicurezza. Io non intendo fare nessuna strumentalizzazione, Ministro, le dico solo che sul nodo di Bologna occorre trovare delle soluzioni strategiche,

e dare finalmente una soluzione strategica a un nodo che non riguarda solo Bologna o l'Emilia-Romagna, ma che riguarda l'Italia e l'Europa. Usiamo tutte le tecnologie, impatto ambientale, la tutela della sicurezza dei cittadini, ma troviamo la forma per fare un ragionamento di merito che sia in grado di dare una risposta vera. Diversamente, ci troveremo sempre in gravissima difficoltà. Confido che questa disponibilità da parte del Governo ci sia e ci saranno la nostra attenzione e la nostra disponibilità a collaborare per trovare una risposta vera a questo gravissimo problema.

Per quanto riguarda la tragedia avvenuta sulle strade della Puglia, credo che quei dodici morti debbano interpellare le coscienze di tutti noi, perché questo è sicuramente il risultato di avere aperto le porte a tutti, per creare, poi, in Italia un nuovo schiavismo, che approfitta di questi disperati, li sfrutta e li costringe a vivere, a lavorare, a muoversi, a essere trasportati in modo disumano. Sostenere che l'Italia ha bisogno di manodopera per poi vedere come la manodopera viene trattata nel nostro Paese, da persone senza scrupoli, per puro motivo di lucro, credo non sia degno di un grande Paese civile, come l'Italia. Il disastro di Bologna interpella le istituzioni, il legislatore, tutti coloro che devono occuparsi della sicurezza sulle nostre strade, sul fatto che ogni giorno circolano centinaia di trasporti pericolosi per gli utenti, per i cittadini, per coloro che sono in viaggio. Anche da questo punto di vista credo che il Ministro abbia ragione, quando dice che non è immaginabile che oggi siano a disposizione avanzati strumenti offerti dalle nuove tecnologie per la guida sicura delle semplici automobili che circolano sulle nostre strade e che questi strumenti non vengano messi a disposizione di mezzi che sono veri e propri ordigni in viaggio. Su questo siamo viaggio. Su questo siamo ben contenti e ben disposti a collaborare. È necessario procedere al più presto, per prevedere che questi mezzi siano dotati di forme avanzate di assistenza alla guida, di dispositivi anticollisione, come ricordava il Ministro, per il controllo della velocità, per la frenata automatica, per il mantenimento automatico della corsia e della distanza di sicurezza; sono tutti strumenti che la tecnologia oggi offre. Noi quindi dobbiamo agevolare, con la legge e con gli incentivi, anche economici, a favore delle aziende che dovranno dotarsene, che ciò avvenga nel modo più rapido possibile. Fermo restando che, comunque, rimane sempre un fattore imponderabile, dovuto al fatto che comunque alla guida di questi automezzi ci sono delle persone, che possono avere un malore o un colpo di sonno. Pertanto, anche da questo punto di vista, Ministro, creo occorra interrogarsi sulla necessità di dotare questi trasporti pericolosi di un secondo autista, come avviene, ad esempio, per i tir che compiono lunghi viaggi. Bisogna anche interrogarsi sulla necessità di prevedere, ad esempio, limitazioni di orario e di giornate. In una giornata da bollino nero, neanche da bollino rosso, c'è da chiedersi se era proprio necessario che questo trasporto dovesse essere effettuato in quell'orario e in quei tempi. Signor Ministro, Fratelli d'Italia e il sottoscritto, come parlamentare dell'Emilia-Romagna, sono certamente pronti a collaborare affinché sulle nostre strade tragedie di questo genere non abbiano più a verificarsi. *(Applausi

anche il Gruppo Partito Democratico si unisce al cordoglio per le famiglie delle persone scomparse ed è vicino alle famiglie e ai feriti

situazioni, sicuramente differenti tra di loro, hanno fatto emergere condizioni molto tragiche su cui sicuramente occorre riflettere. Ringrazio il ministro Toninelli per la puntuale informativa e il presidente Conte per aver trovato le ragioni per potersi recare sui luoghi degli incidenti. Sono due fatti differenti, certamente, perché

di metterci mano e credo che quella sia una legge che il Governo può utilizzare e migliorare. Siamo tutti disponibili a collaborare per trovare le condizioni migliori per applicarla applicarla nel modo più efficace. Da questo punto di vista siamo a disposizione per un confronto assolutamente scevro da strumentalità e focalizzato a trovare

qualsiasi deputato e senatore d'Italia, perché di lì ci passano tutti. Ci passano tutti i cittadini che svolgono un lavoro nel campo dei trasporti o che utilizzano le infrastrutture presenti nel nostro territorio.

Bologna è un nodo assolutamente importante e nevralgico di tutto il Paese: potrebbe parlare un pugliese, così come un senatore valdostano o friulano, perché il nodo di Bologna è il più importante del Paese.

è uno dei motivi per cui noi combattiamo, così seriamente e puntualmente, l'immigrazione clandestina. Quindi, condivido assolutamente la posizione

Per quanto riguarda i fatti di Bologna, abbiamo già detto tanto. Bologna è un nodo strategico. Bene ha fatto il nostro primo ministro Conte a recarsi subito sia a Foggia, che a Bologna.

Vale la pena ricordare, ancora una volta, lo sforzo eroico che tutte le nostre Forze dell'ordine compiono ogni volta che si verificano

Grazie anche per la presenza del Governo sia a Foggia, che a Bologna in un momento terribile per la nazione. Mi permetto di evidenziare

aumento delle nuove tecnologie, ad esempio dei sistemi di frenata, e ciò mal si concilia con una situazione che, in certe zone dell'Italia, è evidente e sotto gli occhi di tutti. Abbiamo le norme per poter prevenire e anche reprimere. Dobbiamo naturalmente effettuare dei controlli. Lei, signor Ministro, questa possibilità ce l'ha.

in chiacchiere. Ora i riflettori si sono accesi su questo problema e su questo dramma, che dovrà necessariamente affrontare anche il problema del trasporto delle merci pericolose, ma che dovrà affrontare il problema del passante. Noi abbiamo sempre indicato il passante Sud. Dobbiamo ricordare, infatti, che l'incidente è avvenuto, sostanzialmente, nel centro di Bologna, nella zona che va dalle due Torri fino alla Madonna di San Luca. È un incidente che ha coinvolto un ristorante, che ha coinvolto strutture pubbliche e che ha portato ad avere 145 feriti, tra i quali, come ricordava proprio lei, signor Ministro, anche undici carabinieri e tre poliziotti. A questo proposito, vorrei, anche a nome del Gruppo Forza Italia, rivolgere un ringraziamento, come avevamo già fatto anche nella giornata di ieri, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, Polizia, ai Carabinieri, ma anche a chi è intervenuto: ai medici e a tutti coloro che negli ospedali si sono fatti carico del senatore Casini)*. Un'organizzazione impeccabile, che si deve naturalmente a quell'amore che gli italiani hanno per il prossimo e anche alla loro competenza. Mi sia consentito di dire, però, che sarebbe anche il momento, dopo tanti anni, di passare dalle parole ai fatti.

realizzare anche questa: avere finalmente un passante a Sud di Bologna per decongestionare quel traffico che in tantissime situazioni, come quella che abbiamo visto ed era sotto gli occhi di tutti, ha portato a quella tragedia immane. Se invece di chiacchierare per tanti anni, di fare convegni, di discutere, fossimo passati realmente dalle parole ai fatti, probabilmente questa tragedia non sarebbe avvenuta.

pronta guarigione. Chiedo, signor Ministro, un impegno da parte del Governo affinché nell'agenda venga inserito questo tema,

risarcimento di quei danni, ma anche ad una soluzione di quell'annoso problema. Speriamo, finalmente, che si possa risolvere.

Una tragedia che ha sconvolto l'intero Paese ma, allo stesso tempo, ha mostrato il volto migliore nel coraggio, nella professionalità e nella solidarietà di tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, dei dei mezzi di soccorso, dei volontari e di tutti i cittadini che nell'immediato degli eventi si sono prodigati per dare un aiuto: questo è il vero volto dell'Italia, costituita da cittadini da sempre uniti nel momento del bisogno. Crediamo che sia necessario trarre una lezione per il futuro da quanto accaduto. Come anche il *premier* Conte ha dichiarato, gli incidenti stradali sono dettati dalla casualità ma, in questo caso, sicuramente ieri c'è stato molto più della casualità. Dobbiamo, non solo chiederci cosa è successo, ma investigare gli eventi e soprattutto proporre in tempi brevi soluzioni che impediscano siffatti accadimenti. Oggi si può disporre di una tecnologia avanzata che può limitare di molto l'errore umano alla guida. Abbiamo e dobbiamo usare la migliore tecnologia a nostra disposizione per impedire morte e distruzione come quella di ieri a Bologna. Contemporaneamente, e al contrario, ieri a Foggia c'è stata una strage di lavoratori stagionali, tutti africani e presumibilmente vittime del caporalato, che lascia veramente sconvolti. Non è possibile che vengano ammassate persone in furgoni senza nessuna dotazione di sicurezza, furgoni assolutamente non idonei al trasporto di persone, lavoratori disperati trattati come se fossero delle cassette di pomodori da portare semplicemente al mercato. È una strage che ci deve interrogare. Nelle zone da cui provengo, nel casertano - pensiamo a Castel Volturno o a Mondragone ogni giorno è possibile vedere questi carri merce stracolmi di vite umane trasportate senza alcuna dignità, per poi essere sfruttate nei campi. È ancora più urgente impedire questo reato che si consuma alla luce del sole, un reato di caporalato che mette a rischio le vite di poveri lavoratori, con caporali che per il loro guadagno mettono a rischio anche la vita di tutti coloro che percorrono le stesse strade di questi furgoni della morte. Mi confortano, quindi, non solo le parole del ministro Toninelli, ma anche quelle del ministro Di Maio, che ieri ha promesso una stretta contro il caporalato e, come ho già detto, le stesse parole di impegno esplicitate dal *premier* Conte. Mi conforta, quindi, che tutto il Governo stia ponendo la massima attenzione e il massimo impegno su criticità diverse, che possono essere foriere di morte e distruzione.

Si capisce perfettamente come la situazione possa essere veramente complicata, non solo per le famiglie in quanto tali, ma proprio per il futuro dei bambini. Avere chiarezza su questo mi sembra determinante anche come fatto di giustizia, per il diritto dei bambini alla famiglia

Sono accaduti in questi giorni dei fatti abbastanza incresciosi. L'interrogazione è stata pubblicata e c'è stata un'incursione che in qualche modo ha privato la Presidente delle volontarie di Croce Rossa di alcune delle prerogative che le spettano in autonomia a norma di legge.

resti in qualche modo confusa. Questa interrogazione è stata presentata contestualmente al Ministero della difesa e al Ministero della salute, da cui dipendono

Credo che potrebbe essere un segnale di buona volontà del Senato che, alla ripresa dei lavori, si cominci proprio dalle interrogazioni, affinché trovino quella risposta che la parola urgenza definisce come dialogo di serenità e, direi, anche di dignità nel rapporto tra senatori e cittadini.

alle 8,15 del mattino del 6 agosto del 1945 gli Stati Uniti sganciarono, sulla città giapponese di Hiroshima, la prima bomba atomica della storia. Il nome della bomba era «Little Boy»; il numero delle vittime dirette non può essere preciso perché molte evaporarono, ma verosimilmente furono tra le 100.000 e le 200.000. Il 10 agosto, tre giorni dopo, su Nagasaki fu lanciato un altro ordigno, «Fat Man». Lo sgancio, però, non fu particolarmente preciso e la bomba brillò in una zona della città difesa dai monti. Nonostante ciò, morirono subito almeno 40.000 persone e molte altre migliaia rimasero ustionate. È davvero difficile pensare cosa abbiano provato quegli uomini e quelle donne che si accingevano ad andare a lavorare o ad accompagnare i bambini a scuola. Non esistevano neppure le immagini di esplosioni atomiche. Nessuno dei cittadini di Hiroshima e Nagasaki aveva visto una tale luce o udito un tale suono così improvviso e devastante. Senza più la città intorno, senza punti di riferimento, in un caldo torrido e colpiti da una forte pioggia radioattiva nera, i sopravvissuti vagarono senza meta. Poi molti, sperando di fermare le terribili scottature, si gettarono nel fiume, che però in alcuni punti ribolliva e ben presto si riempì di cadaveri che galleggiavano. Le bombe atomiche USA furono una prova di forza che gli Stati Uniti volevano manifestare a Mosca. Infatti, già durante il secondo conflitto mondiale si comprese che l'antagonismo futuro sarebbe stato tra le due potenze vincitrice della guerra, USA e URSS. Presidente, cari colleghi, oggi nel mondo ci sono talmente tante armi atomiche che potrebbero far saltare il Pianeta più e più volte. La Russia ha sviluppato un ordigno atomico che si chiama «Satan 2», e ognuna di queste bombe può disintegrare un territorio esteso quanto la Francia. Vorrei ricordare che sul nostro territorio nazionale ci sono armi atomiche statunitensi, le B-61, che ci fanno violare il Trattato di non proliferazione nucleare che abbiamo ratificato nel 1975, oltre a renderci un bersaglio sensibile.

con tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il fenomeno migratorio. Concludo affermando che è fondamentale iniziare un processo di denuclearizzazione e porre fine a quest'economia di guerra, a quel complesso militare industriale paventato da Dwight Eisenower. È giunto il momento di non investire più in strumenti di morte, ma in cultura della vita.

Come ricordava il Ministro poco fa, a Foggia, in soli tre giorni, in due distinti incidenti stradali, hanno perso la vita sedici braccianti agricoli, che tornavano dal lavoro nei campi. Apprezzo molto la risposta del Ministro di oggi e appezzo anche che il presidente Conte e il ministro Salvini siano stati oggi a Foggia per poter subito intervenire sul tema della lotta al caporalato. Ciò detto, il 9 agosto dello scorso anno, a San Marco in Lamis si è verificato un tragico evento, una strage di mafia, in cui hanno perso la vita anche due cittadini innocenti, i fratelli Luciani, testimoni oculari di un agguato mafioso. Dopodomani ricorre il primo anniversario di questo tragico evento, e i fratelli Luciani saranno ricordati a San Marco in Lamis con vari eventi commemorativi. Oggi, oltre a unirmi al giusto e doveroso ricordo, voglio ancora una volta richiamare l'attenzione di quest'Assemblea e del Governo rispetto al gravissimo problema rappresentato dalla quarta mafia italiana, ovvero le mafie della della provincia di Foggia, come sono state definite dall'ex procuratore nazionale antimafia. In questa occasione oggi voglio ribadire l'assoluta necessità che si intensifichino tutte le azioni di contrasto che il nostro ordinamento prevede, a partire dall'aumento delle Forze dell'ordine, per finire all'aumento dei presidi giudiziari. A quest'ultimo proposito, ritengo non più rinviabile l'istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia, al fine di aumentare la qualità e la quantità delle indagini antimafia. Su questa necessità si è espresso nell'ambito delle risoluzioni sulle mafie foggiane del 18 ottobre 2017, e su tale aspetto ho appena presentato un disegno di legge. Concludo ricordando ancora i fratelli Luciani e tutte le altre vittime di mafia, e voglio aggiungere che noi tutti, in quest'Aula e fuori, non ci arrenderemo finché le mafie non saranno sconfitte. E noi alla mafia diciamo questo: non ci arrenderemo mai!

Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio porre l'attenzione di questa Assemblea sulla situazione della sanità nel mio collegio di elezione nelle Marche, che comprende la provincia di Ascoli Piceno, come tutti voi sapete, tristemente colpita dagli eventi sismici del 2016 che sono stati oggetto di recenti lavori legislativi svolti anche da questa Assemblea e a cui ho avuto l'onore di partecipare. Data quindi la delicatezza e l'importanza del tema in questione, occorre parlare chiaro, perché non si può giocare sulla salute e l'assistenza sanitaria pubblica, come sta facendo adesso la Regione Marche, le cui scelte risultano sempre più irrazionali, soprattutto nella zona Sud della nostra Regione. È della settimana scorsa, infatti, la votazione della conferenza dei sindaci della provincia di Ascoli Piceno che, in spregio al principio di rappresentatività della popolazione e seguendo pedissequamente le direttive regionali, avallato la scelta della Regione Marche di costruire un nuovo ospedale lontano dai due centri principali della provincia, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che vedranno, quindi, i loro attuali ospedali, già oggetto di pesanti tagli nel corso degli anni (in particolar modo quello di San Benedetto del Tronto), ridursi nei fatti a essere dei presidi ospedalieri, nell'attesa che si realizzi, magari tra qualche decennio, un nuovo ospedale di primo livello, guarda caso in una realtà comunale amministrata da una lista civica riferibile all'area politica di chi attualmente governa la Regione e che andrà al rinnovo delle cariche comunali il prossimo anno. Su queste scelte resta il dubbio se esse siano dettate siano dettate da un disdicevole opportunismo politico e completamente sganciate dal diritto alla salute che la Repubblica garantisce costituzionalmente ad ogni cittadino. Ora la vera domanda da porsi è: cosa accadrà alla sanità nel Piceno? In attesa di questo fantomatico ospedale unico della Provincia, di cui non si hanno ancora un progetto e un *iter* certo di lavori e la cui collocazione è stata decisa da un algoritmo, che servizi erogheranno gli attuali ospedali di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto? Che visione politica ha la Regione Marche? Tale Regione, invece di rafforzare alcuni servizi essenziali come quelli sanitari nella sua zona (la più colpita dai recenti eventi sismici), nei fatti attua un ridimensionamento dell'esistente e propone miraggi di ospedali unici, con evidenti mire elettorali di breve periodo. Essa applica, inoltre, in maniera opportunistica le previsioni normative del decreto Balduzzi, relative ai bacini di utenza ospedalieri, parametrando detti bacini di utenza, solo in base ai confini regionali, in un'area di confine della Regione che, come nel caso di San Benedetto del Tronto, serve anche gran parte dell'area Nord del confinante Abruzzo? In conclusione, mi sembrava doveroso porre l'attenzione di tutti voi su queste scelte della Regione Marche, che stanno andando anche contro gli sforzi che questa Assemblea ha svolto e continuerà a svolgere per far rinascere i luoghi colpiti dal terremoto del 2016, sia quelli colpiti direttamente, come la zona montana dell'Ascolano, sia quelli colpiti indirettamente nel loro principale volano economico, il turismo, come nel caso della zona della Riviera delle Palme in cui insiste l'attuale ospedale di San Benedetto del Tronto.

E quando scendi la prima volta il cuore ti sale in gola, anche lo stomaco a dire il vero. La prima volta che si scende in miniera si vomita. Quando l'ascensore parte, si sente come uno scoppio, poi ci fai l'abitudine. Ma la prima volta pensi che qualcosa sia andato storto, che stai precipitando, che l'ascensore sta scendendo troppo velocemente. Tutto diventa buio e quelle poche luci che vedi ad intermittenza ti fanno scoppiare la testa, tanto che preferisci chiudere gli occhi. di un passaggio di uno spettacolo teatrale di un giovane catanese, Alessandro Idonea che, prendendo spunto dalla strage di Marcinelle, ha scritto questo pezzo: «262 vestiti appesi». Furono appunto 262 quei vestiti che non furono reindossati dai loro titolari; 262, spesso giovanissimi, stranieri per la maggior parte; 136 di loro, italiani.

Credo sia importante ricordare in queste Aule questa strage proprio oggi, immediatamente dopo l'informativa del Governo, che ci ha ricordato, ancora una volta, la strage di ieri di nuovi cittadini stranieri, morti per esempio in Puglia. Credo sia di monito a tutti noi non soltanto per ricordare il sacrificio di quei nostri concittadini, ma anche per indurci a continuare nella nostra battaglia per aumentare e migliorare i livelli *standard* di sicurezza sul lavoro e anche per tenere presente che quei migranti e quei braccianti, che anche solo poche ore fa sono deceduti, non sono altro che la proiezione oggi dei nostri concittadini di allora che, a partire dagli anni Cinquanta, lasciarono il nostro Paese in cerca di condizioni migliori. *(Applausi).* Nell'augurare a tutti, a quelli che ci sono e anche a quelli che ormai sono andati via, una buona vacanza, comunico che le Commissioni riprenderanno i propri lavori da martedì 4 settembre. Le Commissioni sono comunque autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.